cui risponderà il ministro delle comunicazioni, onorevole Gentiloni. Ricordo ai colleghi che un senatore per ciascun Gruppo potrà rivolgere domande al Ministro per non più di due minuti, e sottolineo due. Il Ministro risponderà congiuntamente a tutte le domande per non più di dieci minuti. Ciascun interrogante potrà successivamente replicare per non più di un minuto.

sarebbe stato opportuno un provvedimento che non riguardasse solo la dottoressa Bergamini, ma tutte le persone coinvolte.

non so se lei ascolta e vede i servizi parlamentari

me ne sono andato l'8 febbraio 2001, pochi mesi prima delle elezioni politiche. Io non volevo una RAI schierata prima delle urne, convinto com'ero che l'equilibrio avrebbe giovato anche al centro-sinistra. Vidi invece un grande attivismo di Zaccaria che convocava direttori e autori di programmi. Mandai uno, due, tre segnali. Poi me ne andai. In seguito accadde ciò che sappiamo: i programmi Travaglio-Luttazzi, i casi Santoro, una Rai schieratissima». C'è, dunque, la RAI dei manganellatori mediatici, dello squadrismo

RAI-Mediaset Alleanza Nazionale ha apprezzato la solerzia con cui la RAI ha attivato l'indagine interna e, fiduciosa, attende. Tuttavia, prima di assumere eventuali provvedimenti ambigui come quello odierno, non era forse meglio attendere l'esito finale di quest'indagine? Secondo quesito. Proprio ieri la maggioranza che regge questo Governo ha deciso di accelerare la discussione del disegno di legge sulla *governance* RAI, infischiandosene delle argomentazioni avanzate dal centro-destra che, glielo garantisco, signor La situazione del futuro RAI è abbastanza confusa: una parte della sua maggioranza la vorrebbe privatizzata, un'altra, invece, non ci sente proprio da questo punto di vista. Veltroni ha proposto la figura dell'amministratore unico, di fatto sconfessandola, signor Ministro, perché lei invece vuole una pletora di personaggi, addirittura undici, nel consiglio di amministrazione della fondazione RAI e poi altri 5 nel consiglio di amministrazione della RAI. allora, signor Ministro, nel paese delle meraviglie, in cui lei vive con Alice (beata ingenuità), siete davvero convinti che questo provvedimento possa rilanciare la RAI e allontanare i partiti? Terzo ed ultimo quesito. Lei purtroppo ha condiviso l'arroganza con cui il ministro dell'economia Padoa-Schioppa ha revocato il professor Petroni dal consiglio di amministrazione della RAI per sostituirlo con un uomo di stretta osservanza prodiana. Dopo la sentenza del TAR, che ha reintegrato Petroni, le chiedo: crede opportuno continuare sulla strada della tracotanza del ministro Padoa-Schioppa? Non ritiene utile, al contrario, anche per rasserenare il clima, chiedere le dimissioni del presidente abusivo Petruccioli, che lei sa essere stato senatore della sinistra, oltretutto sfiduciato dalla Commissione di vigilanza RAI e quindi dal Parlamento? [RUSSO

degli assetti democratici di un Paese, di che cosa i cittadini e le cittadine debbano sapere, di come debbano saperlo, se devono, in definitiva, essere o meno informati. A me pare che a questo alludano gli intrecci fra strutture RAI e Mediaset emersi negli ultimi tempi, il passaggio di donne e uomini da un'azienda all'altra, come se la specificità del servizio pubblico, la sua filosofia, la sua missione non comportassero una scelta professionale specifica. Si è parlato su un giornale importante, «la Repubblica», di una struttura occulta. comunque, che stiamo parlando di una rete di interessi occulti nelle mani di Berlusconi, tesi a consolidare una trama di interessi economici e personali, che a volte utilizzano la politica per finalità di profitto individuale o di azienda e che creano un sistema di valori a livello popolare che tiene nascoste in un cono d'ombra le inchieste sociali, le sofferenze della popolazione, le condizioni in cui vivono lavoratori, pensionati, donne, giovani, precari. Insomma, un servizio pubblico che rischia di essere al carro della mercificazione privata e di non svolgere più alcuna funzione. Credo che sia che sia importante che il Governo svolga un ruolo fondamentale per il rilancio del servizio pubblico ed è per questo che le chiedo, signor Ministro, quali procedure parlamentari

signor Ministro, mentre si discute e si favoleggia in buona parte di intercettazioni, la RAI è in una condizione di sostanziale paralisi, che non le impedisce, tuttavia, come hanno pubblicato i giornali nelle ultime giornate, di fornire un'informazione sbilanciata a favore della maggioranza e del Governo. È in atto ancora una sorta di accanimento per cercare di tenere lontano dal consiglio di amministrazione della RAI il consigliere Petroni, nonostante una sentenza della magistratura confermi che non vi siano state motivazioni né politiche, né, soprattutto, di legittimità giuridica per operare quella scelta. Vi è poi - lo ricordo - una sfiducia formale della Commissione di vigilanza nei confronti del presidente dell'Azienda Petruccioli, perché è venuta meno - questa è la motivazione - una sostanziale condizione di garanzia e di equilibrio, che doveva invece essere alla base di un assetto complessivo della RAI. Alla luce di tutto questo le chiedo

Soprattutto, come esponente dell'UDC, partito che ha espresso la disponibilità a dialogare, mi interessa sapere se vi è da parte sua e del Governo la disponibilità ad accettare modifiche ai provvedimenti legislativi che sono in essere nei due rami del Parlamento per una riforma complessiva della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

ancor più gravi appaiono le prospettive future, con un aumento incontrollato dell'indebitamento. In qualche modo la RAI sembra essere un doppione fedele di Alitalia, con gli stessi identici problemi: un numero spropositato di dipendenti, assunti in gran parte con dinamiche clientelari, una gestione decisamente "romanocentrica", malgrado il 70 per cento di economia reale passi nelle Regioni padane del Paese, che dovrebbero essere ben diversamente valorizzate in termini di gestione e strategia aziendale. A fronte di questa situazione, non si intravede nessun disegno strategico per invertire la tendenza negativa e riportare l'Azienda televisiva sulla strada di un futuro certo e adeguato alle esigenze dell'informazione pubblica. Abbiamo inoltre assistito a situazioni paradossali, come tutto l'affare del consigliere Petroni, sostituito dal ministro Padoa-Schioppa con atto d'imperio e reintegrato d'ufficio dal TAR del Lazio. Lo stesso Ministro aveva descritto in Commissione vigilanza il dottor Petroni come individuo inaffidabile e come unico responsabile della crisi aziendale RAI. Si chiede quindi di conoscere come finirà la questione Petroni, se al ministro Padoa-Schioppa, come succederebbe in qualunque Paese normale, oltre alle dovute dimissioni, visto che non è la prima figuraccia che fa (ricordiamo la Guardia di finanza), sarà richiesto anche il risarcimento economico per tutta la faccenda e soprattutto quali siano le linee strategiche aziendali per il rilancio della RAI, o se più semplicemente i cittadini dovranno continuare a pagare il canone per vedere telegiornali che sembrano l'ufficio stampa del Governo o programmi d'intrattenimento con attempati artisti pagati centinaia di migliaia di euro per fare in diretta TV *spot* pubblicitari al presidente Prodi.

signor Ministro, il contratto di servizio tra lo Stato e la RAI, al quale il suo Ministero sovrintende, obbliga la RAI a fornire un'informazione completa, obiettiva, imparziale e conforme ai princìpi costituzionali del pluralismo informativo. Per l'informazione politica della RAI - mi spiace dire questo - ciò non è rispettato. In particolare, per i servizi radiofonici di «GrParlamento» e per quelli televisivi dei servizi parlamentari si raggiungono livelli record di invadenza partitica, ma ciò è vero anche per le altre testate giornalistiche maggiori. La lottizzazione partitica delle redazioni a tutto vantaggio dei partiti maggiori dei due schieramenti è evidente; lo spazio riservato ad essi è straripante e le iniziative dei partiti maggiori vengono diffuse come contributi alla partecipazione civile e democratica. Talora, e per fortuna solo talora, gli stessi fatti vengono manipolati per trarne vantaggi partitici e questo coinvolge la deontologia professionale di importanti responsabili dell'informazione radiofonica e televisiva, come testimoniano le recenti intercettazioni telefoniche che descrivono una commistione tra testate della RAI e di Mediaset per addomesticare fatti politici sconvenienti per una parte, commistione che è contraria ai princìpi del pluralismo televisivo e a quelli della concorrenza. Le chiedo, signor Ministro, cosa intenda fare, con la massima tempestività, per ricondurre subito nel loro alveo proprio i servizi radiofonici e televisivi parlamentari e, più in generale, per allontanare quanto sia più possibile l'ingerenza dei partiti sulla RAI, restituendo alla RAI credibilità,

dopo la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche tra dirigenti RAI e Fininvest, non più sottoposte a segreto, molti hanno osservato che erano cose risapute, alcuni hanno persino detto che bisognava minimizzare perché non era successo nulla. Erano certo cose risapute, ma non di tale gravità, anche se ormai una parte dell'opinione pubblica aveva digerito l'anomalia delle immissioni in RAI di ex dirigenti Fininvest come un fatto scontato, anche se non naturale o motivato. A me pare che le intercettazioni abbiano messo in evidenza un vero spionaggio industriale, organizzato in modo eccellente, cioè una sorta di catena di comando. L'obiettivo, come si è visto, era manipolare l'informazione a favore dell'allora capo del Governo. Una catena organizzata pagata dai contribuenti. L'organigramma era molto articolato, una gerarchia che occupava le caselle strategiche: le direzioni, le reti, i telegiornali. Non è il duopolio, ma una sorta di monopolio molto articolato,

agli interessi del momento e che non si faccia distrarre dalle politiche del momento e dalle contingenze, come, per esempio, la ricerca di un accordo sulle riforme elettorali e costituzionali.

signor Ministro, la finanziaria 2008, in corso di approvazione, equipara, per alcune disposizioni attinenti il trattamento economico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai dipendenti delle società partecipate o a prevalente partecipazione pubblica. Tuttavia, è stata volontariamente esclusa tale equiparazione per i professionisti che operano nei servizi della RAI, i quali intrattengono rapporti di lavoro tramite contratti di prestazione. Una equiparazione economica avrebbe potuto consentire, in futuro, una estensione dell'applicazione della normativa che regola la cosiddetta responsabilità amministrativa. Questa, come lei ben sa, signor Ministro, è quella speciale responsabilità che obbliga personalmente il pubblico funzionario, il pubblico amministratore e, in generale, il pubblico agente a risarcire i danni eventualmente causati all'erario per effetto di comportamenti dolosi, o almeno gravemente colposi, attuati nell'esercizio delle funzioni e in violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni di servizio. A mio avviso, infatti, un professionista che stipula un contratto con la RAI società partecipata pubblica, ricordiamolo - ha il dovere di rispettare le norme dettate per garantire l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici. Sappiamo che, qualora queste norme siano violate, è la RAI a dover sopportare la sanzione comminata dall'Autorità garante e saranno i soldi dei cittadini, versati tramite il canone, a dover essere spesi per sopperire alla mancanza di professionalità di questi pseudoprofessionisti che abusano dell'influenza loro concessa dal mezzo Chiedo quindi, Ministro, se non sia giunta l'ora di predisporre una normativa che obblighi la RAI a rivalersi per i danni subiti, sia a livello di immagine che a livello monetario, su questi professionisti, obbligando la stessa a rescindere loro il contratto per uso improprio del mezzo televisivo.

considerate le vicende relative all'Azienda che gestisce il nostro servizio pubblico radiotelevisivo, da quella più recente delle intercettazioni, che hanno fatto emergere il clima collusivo che permeava RAI e Mediaset, a quella che oramai da mesi pende presso i tribunali, ossia la «nomina Fabiani-revoca Petroni», che oggi è divenuta «restauro Petroni-sospensione Fabiani»; considerato che l'ultima tra le vicende menzionate ha soltanto riaperto la problematica della rottura dell'accordo istituzionale tra maggioranza e opposizione, avvenuta con la nomina di un presidente, quale figura di garanzia, espressione della maggioranza, anziché dell'opposizione, quali iniziative intende assumere il Governo per porre fine a questo stato di immobilismo decisionale, che impedisce all'Azienda di rispondere alla sua missione di fornire un servizio pubblico che garantisca il principio del pluralismo

Signor Presidente, cercherò di rispondere ai diversi quesiti posti dagli onorevoli senatori, molti dei quali riguardano la natura e le la natura e le conseguenze di un fatto accaduto la scorsa settimana, cioè l'inchiesta pubblicata da «la Repubblica» riguardo ai rapporti RAI-Mediaset nel 2005. Credo che la RAI abbia fatto bene a non minimizzare gli episodi che emergevano da quell'inchiesta.

ad incaricare i servizi giuridici e legali dell'Azienda di costituirsi parte offesa, al fine di interloquire direttamente con gli uffici giudiziari e al fine di attivarsi per acquisire, se disponibili, le trascrizioni delle intercettazioni apparse sui giornali e di eventuali altre. Voi sapete che proprio oggi, in relazione a questa attività, la RAI ha deciso di sospendere un suo dirigente, la dottoressa Deborah Bergamini; non si è trattato di un provvedimento disciplinare, ma di una sospensione, per così dire, cautelare, in modo da consentire al comitato etico di completare gli accertamenti e alla stessa dottoressa Bergamini di chiarire al meglio la sua posizione. Naturalmente, non si tratta di un caso singolo e certamente il Governo non ha alcun titolo ed alcun elemento per esprimere giudizi su casi singoli. Non si tratta di cercare capri espiatori. Penso che sia una attività d'inchiesta interna che la RAI ha tutto il diritto e, direi, il dovere di svolgere in piena autonomia, perché credo che quanto è emerso da quella inchiesta giornalistica sia piuttosto grave. Emergeva, cioè, un clima collusivo, che faceva riferimento anche ad un problema di natura politica sul quale, invece, certo il Governo può esprimere la sua opinione: opinione: non si trattava semplicemente di contatti tra due aziende concorrenti, come la Coca Cola e la Pepsi Cola, ma di contatti tra due aziende televisive che, secondo questa inchiesta giornalistica che giustamente è importante acclarare e accertare, sembravano tesi anche, ad esempio, a presentare in un certo modo, con una certa tempistica i risultati delle elezioni regionali del 2005: quindi, questioni che hanno a che fare con l'interesse del Parlamento al pluralismo e alla corretta rappresentazione dei fatti. Credo di poter tranquillizzare, da questo punto di vista, il senatore Ripamonti sul fatto che l'intenzione del Governo non solo alla luce di questi fatti ma come suo indirizzo - quale che sia l'andamento del dialogo tra le forze politiche sulle regole e sulle leggi elettorali è di portare avanti i suoi disegni di legge, depositati in Parlamento, sia sul sistema televisivo che sul conflitto di interessi. Molti dei senatori interroganti hanno chiesto cosa intenda fare il Governo per cercare di far uscire dalla sua situazione di instabilità e di difficoltà la televisione pubblica, la RAI. RAI. Credo che il Governo abbia una risposta semplice, anche se naturalmente soggetta a discussione parlamentare: la nostra risposta semplice è nel disegno di legge che il Governo ha proposto al Parlamento e in particolare al Senato.

c'è l'evidenza in tutta l'opinione pubblica della necessità di provvedere con urgenza a risolvere un problema che si trascina da quindici da quando un cambio di sistema politico nel nostro Paese ha prodotto una sorta di instabilità permanente nella televisione pubblica che oggi non è più sostenibile.

Gli obiettivi sono semplici a dirsi e molto difficili - spero non sia veramente Alice nel paese delle meraviglie - da attuarsi e sono quelli di dare più autonomia dal Governo e dai partiti, e più capacità di decisione all'Azienda. Oggi la RAI, purtroppo, è un'azienda in cui per decidere qualunque cosa i processi sono incredibilmente lenti. D'altro canto, la tradizionale dipendenza dai partiti, una volta passati dal sistema della prima Repubblica ad un sistema bipolare, provoca tendenze continuamente oscillanti, che destabilizzano l'Azienda e possono costituire un pericolo e una minaccia per il pluralismo. Il Governo, con gli strumenti a sua disposizione, che sono ‑ come ricordava il senatore Paolo Brutti ‑ quelli dell'indirizzo, del contratto di servizio, della verifica dell'attuazione, è pronto ad intervenire senza sovrapporsi alle competenze della Commissione di vigilanza, naturalmente, ma cercando, di fronte a fatti gravi, di esprimersi per far rispettare i princìpi contenuti nel contratto di servizio. Per quanto riguarda le vicende più interne al consiglio di amministrazione, al rapporto tra i vertici aziendali e l'azionista, credo che a chi ha chiesto una previsione su cosa farà il Governo, su come andrà a finire la vicenda si tratta di dare semplicemente due risposte: la vicenda di merito si concluderà il prossimo 4 dicembre di fronte alla IV Sezione del Consiglio di Stato, alla quale il Ministero dell'economia ha fatto ricorso chiedendo una istanza sospensiva della delibera del TAR; dal punto di vista generale, considero questa - ahimè - una ulteriore tappa di una storia che va avanti da molti anni. Prima il senatore Novi ricordava una intervista di Pierluigi Celli, che è stato uno dei protagonisti di questi anni; la realtà è che da quattordici o quindici anni abbiamo una azienda di servizio pubblico continuamente destabilizzata da una situazione alla quale bisogna porre rimedio con una riforma. Nei cinque anni di Governo di centro-destra a ciò si è aggiunto il problema che in gergo chiamiamo «conflitto di interessi», cioè il fatto che il Presidente del Consiglio era anche il proprietario di televisioni commerciali. La crisi della RAI, però, era nata prima ed è continuata dopo e per porvi rimedio non c'è altra strada, credo, se non una riforma come quella che il Governo ha presentato e sulla quale il Senato ha il diritto e - io ritengo - il dovere di esprimersi con proposte di modifica, di correzione e, se possibile, di miglioramento. Infine, signor Presidente, sono state poste un paio di questioni che esulavano da quelle più direttamente riguardanti i rapporti RAI-Mediaset, le inchieste in corso, il progetto di riforma del Governo ed altro. Con riguardo al funzionamento della testata parlamentare,

Quindi il Governo può essere attivato - e certamente in base a questa segnalazione si attiverà - per verificare che il rapporto con le Presidenze di Camera e Senato e l'obiettivo di potenziamento vengano realizzati. Per quanto riguarda problemi più relativi agli equilibri tra le diverse forze politiche (temi su cui sono intervenuti in diversi, ad esempio il senatore Paolo Brutti e il senatore Novi), è chiaro che è soprattutto la Commissione di vigilanza che deve attivarsi, ma certamente il Governo si riserva di intervenire, se vi fossero violazioni tali da mettere in discussione i fondamenti del contratto di servizio. Il senatore Cutrufo posto un quesito relativo all'articolo 144 della legge finanziaria 2008, che fissa un tetto ai compensi per le aziende partecipate dallo Stato che non sono quotate in Borsa. Se, da

in un regime di competizione nel quale la RAI inevitabilmente è inserita, che si possa imporre un trattamento completamente diverso per la televisione pubblica rispetto alle televisioni commerciali.

quale che sia la sorte dell'articolo 144 della legge finanziaria 2008, il principio di responsabilità amministrativa sussiste comunque. Anche negli ultimi mesi, per

di responsabilità, com'è giusto che sia in un'azienda pubblica.

con le intercettazioni telefoniche. Rimango altrettanto convinto che il provvedimento cautelativo emanato da parte della RAI nei confronti di un dirigente dovrebbe essere esteso anche a tutti gli altri; comunque, speriamo di andare in questo senso.

l'*Authority* per le telecomunicazioni, per quanto riguarda il TG1 e tutta l'informazione RAI ha sostenuto, affermato e certificato che era molto più equilibrata l'informazione RAI del del tempo di Berlusconi nell'aprile del 2005 di quella dell'aprile 2007. Voglio ricordare che il TG1 diretto dal dottor Riotta dà a Prodi il doppio del tempo che gli dedicava il Voglio anche ricordare che la dottoressa Bergamini è stata sospesa probabilmente perché conosce tre lingue, che parla correntemente, è laureata in lettere con il massimo dei voti, ha conseguito un dottorato negli Stati Uniti, ha lavorato per la catena Bloomberg dal 1997 al 1999 è stata capo redattore di un *network* di informazione economica a Parigi. Sostanzialmente, presenta qualità ed un *curriculum* che è raro riscontrare tra i dirigenti RAI: per questo l'avete sospesa.

Se in RAI non entra la pubblicità, vi dovrete rifare - come siete soliti, ovviamente - sulle tasche dei cittadini. Con cosa? Con l'odioso canone. E allora, anche qui, non avete fatto nulla per combattere l'evasione, ormai arrivata

penso che dobbiamo interessarci a fondo del tema della pubblicità, ma in maniera completamente diversa e alternativa rispetto a come veniva detto poco fa. È vero che la pubblicità sta imponendo una distorsione e un condizionamento della qualità del prodotto televisivo. Se, infatti, l'inserzione pubblicitaria sceglie la *soap opera* o «L'Isola dei famosi» come paradigma del rapporto fra mercato e qualità per rivolgersi ad un pubblico di massa, la qualità crolla. Il servizio pubblico deve anche porsi il problema e avere la forza e l'autorevolezza di governare, regolamentare, programmare,

egemonia culturale, produzione di contenuti, costruzione di senso comune, tecnologia e grande professionalità dei giornalisti. A ciò devono tendere le riforme che con questo Governo e questa maggioranza dovremmo fare.

del ministro Padoa-Schioppa ha generato la crisi nel consiglio d'amministrazione e, di conseguenza, in Commissione di vigilanza. È una contraddizione con la quale, a mio avviso, dovete fare i conti. Sono parzialmente soddisfatto per la conferma dell'apertura e della disponibilità al dialogo sulle riforme con l'opposizione. L'invito dell'UDC è a non perdere un'occasione, che potrebbe portare ad un rinnovamento sostanziale, tenendo separato il controllo istituzionale sulla RAI, che è sacrosanto, dal controllo dei partiti, che è una forma di degenerazione che va respinta. Non sprechiamo questa occasione; no a logiche punitive nella riforma del servizio pubblico e, soprattutto, come ultima considerazione, l'accettazione di qualche suggerimento sul fronte della privatizzazione della RAI, che probabilmente è un elemento risolutivo, più che lo spezzettamento che in qualche caso si intravede nei provvedimenti al nostro esame.

mantenuto dal canone pagato dai cittadini, soprattutto padani, anche se lei si è ben guardato dal ricordarlo. Basti dire che la sola città di Varese, con 85.000 abitanti (come attestano dati di qualche settimana fa), paga più canone di tutta la città di Napoli, che è dieci volte più grande. Quindi, se vuole veramente rendere un servizio al Paese, faccia una sola riforma: mantenga qualche sede regionale per l'informazione locale e venda tutto il resto a qualche privato, magari arabo, visto che hanno i soldi e sono vostri amici, così almeno i giornalisti strapagati, schierati e faziosi, ma dal cognome nobile e famoso, ed i vari Celentano e Benigni, per i loro *spot* a Prodi, li pagherà qualcun'altro. di due, senatore Galli. GALLI *(LNP)*. Non entro nel merito, ma credo che anche lei convenga con noi che se togliessimo, con rispetto per tutti, i raccomandati, i parenti, gli uomini di partito e tutto il resto, alla RAI resterebbero ben in pochi.

Ministro, la ringrazio e mi dichiaro soddisfatto per le osservazioni che ha voluto fare. Spero proprio che le sue parole relative ai servizi parlamentari abbiano un seguito immediato, perché ne sentiamo proprio l'esigenza. La mancanza di imparzialità di questi servizi è evidente a tutti. Le confermo qui l'impegno mio personale e del mio Gruppo sulla legge in discussione al Senato, perché anch'io penso che essa sia lo strumento principale per portare la RAI fuori dall'influenza dei partiti.

provi ad affrontare il problema della sostituzione del canone con il passaggio al carico fiscale del mantenimento e del pagamento dei servizi radiotelevisivi. sono parzialmente soddisfatto per la risposta e soddisfatto per la premessa. In due parole, ritengo che il Governo abbia fatto bene a valutare il problema delle intercettazioni come fatto molto grave, lo scambio di informazioni e di valutazioni di scelte editoriali mi pare fosse teso a manipolare l'informazione a favore dell'allora Capo del Governo. Queste valutazioni mi soddisfano. Sono parzialmente soddisfatto relativamente alla risposta sul conflitto di interessi: non tanto sul fatto che il Governo abbia dichiarato apertamente che questo non sarà posto sul piatto della bilancia di un'eventuale trattativa politica, quanto per il fatto che, dal momento che si è trattato di un vero monopolio incardinato su un colossale conflitto di interessi, bisogna tentare di indicare dei tempi. Certo, ciò non dipende solo dal Governo, ma anche dal Parlamento. Però, il Governo deve legittimamente indicare i propri obiettivi. In ogni caso,

e proponevo di emanare una normativa per evitarla. Chi decide di candidarsi non farà più il mestiere di giornalista, così come il magistrato che si candida non farà più il magistrato. È normale, perché esiste un vincolo oggettivo di interesse privato tra questi signori e la politica del Paese.

dovrebbero avere il coraggio di rassegnare le dimissioni e consentire una ricomposizione del vertice, rispettosa dell'asse istituzionale in base al quale

contro il teppismo e la violenza negli stadi e l'appello alle tifoserie affinché sia bandita ogni forma di violenza negli stadi, anche a difesa della Polizia di Stato, custode della nostra sicurezza.